Mutuo un'espressione di un mio predecessore. la Conferenza dei Capigruppo riunitasi questa mattina ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori per le prossime due settimane, fino a giovedì 29 gennaio. In relazione ai lavori tuttora in corso presso le Commissioni riunite la, 5a e 6a sul disegno di legge collegato recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale - già all'ordine del giorno di oggi la settimana corrente sarà dedicata al seguito della discussione del disegno di legge sulla sicurezza pubblica. Oggi pomeriggio si svolgeranno le sole repliche dei relatori e del Governo. Sarà quindi tolta la seduta per dare tempo ai Gruppi di presentare eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dal Governo. Il termine per i subemendamenti è stato fissato alle ore 20 di questa sera. Pertanto l'esame degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge avrà inizio a partire dalla seduta antimeridiana di domani. In apertura della seduta pomeridiana di domani, la Presidenza ricorderà il novantesimo compleanno del senatore a vita Giulio Andreotti. Successivamente potranno intervenire i Gruppi per 5 minuti ciascuno. Gli orari delle sedute di questa settimana sono stati ridotti per consentire più ampi spazi di attività alle Commissioni, che avranno a disposizione anche 1'intero pomeriggio di giovedì prossimo, in particolare per l'esame del disegno di legge sul federalismo fiscale, nonché dei decreti-legge presentati al Senato. L'inizio della discussione da parte dell'Assemblea del disegno di legge sul federalismo fiscale è stato stabilito per le ore 11 di martedì 20 gennaio. Tutta la prossima settimana sarà quindi dedicata alla trattazione di tale argomento, per la quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi secondo lo schema riportato in allegato al calendario dei lavori. A partire dalle ore 15 di lunedì 26 gennaio e fino alla seduta antimeridiana di mercoledì 28 (data della scadenza), è prevista la discussione del decreto-legge recante misure anticrisi, al momento all'esame della Camera dei deputati. La ripartizione dei tempi sarà successivamente stabilita. Nella seduta pomeridiana di mercoledì 28 gennaio si svolgeranno la Relazione del Ministro della giustizia sullo stato della giustizia e il conseguente dibattito, previa ripartizione dei tempi tra i Gruppi secondo la prassi. La discussione del documento della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata nella Circoscrizione Estero avrà invece luogo, in relazione al differimento dell'esame del federalismo fiscale, nella seduta antimeridiana di giovedì 29 gennaio. Seguirà l'eventuale seguito di argomenti non conclusi. Il sindacato ispettivo tornerà a svolgersi nella seduta pomeridiana di giovedì 29 gennaio. Ove la discussione del disegno di legge sulla sicurezza non dovesse concludersi entro i termini del calendario, l'esame riprenderà nella giornata di martedì 3 febbraio. In relazione ai numerosi provvedimenti previsti dal calendario corrente, la calendarizzazione degli altri argomenti sollecitati dai Gruppi e dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sarà presa in considerazione in una prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo.

quindi illustrare le motivazioni che ci hanno portato a questa decisione. ovviamente di una motivazione tutta politica, e non tecnica, che manifesta uno stato di disagio da parte del mio Gruppo; Gruppo; disagio che nasce dal fatto che quest'Aula deve sempre esaminare, in tutta fretta e con una straordinaria compressione dei tempi, una decretazione d'urgenza che è stata l'unica che ha occupato i lavori del Senato, ovviamente se si fa eccezione per il famoso lodo Alfano. anche la schizofrenia con cui si accelerano e si interrompono i lavori: penso, ad esempio, al disegno di legge sulla sicurezza

continueremo ad esaminarlo ancora nel prossimo mese. Non mi pare che nell'economia e nell'omogeneità dei lavori parlamentari questo sia un indirizzo del tutto lineare.

Grazie, Presidente.

provvedimento lo discuteremo a febbraio, qual è il motivo di una compressione a poche ore per la presentazione dei subemendamenti? Mi pare che questo sia un modo

una materia ed un campo in cui il mio Gruppo ha lavorato con serietà e tenacia, non risparmiandosi neppure durante il

più serrata, perché abbiamo parlato di lavorare il lunedì, piuttosto che il venerdì, ma ancora non abbiamo dati significativi e concreti sul tema. Non vogliamo disertare le Aule, ma starci dentro.

maniera più severa possibile. Mi perdoneranno i colleghi, ma se qualcuno di noi - e ci mettiamo tutti dentro - non è presente in Aula,

o tre giorni), ancorché si riesca a modificare il Regolamento sul tema, bisognerà probabilmente arrivare alla stessa determinazione assunta dalla Camera dei deputati,

senza ferie o pause, ma con tempi che consentano a chi è oggi opposizione - e speriamo

non dialogando e parlando di confronto, ma dando tempi giusti in Parlamento, perché il confronto deve avvenire nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari.

ha sfiorato quest'ipotesi inserendola nel contesto di un ragionamento molto più ampio. Sta a me constatare e dare atto di come la vostra partecipazione e il vostro contributo al dibattito parlamentare in questa legislatura sia stato, non soltanto corretto, ma composto e denso di propri contenuti, poi condivisibili o meno non non ho mai assistito ad atteggiamenti ostruzionistici, anzi a comportamenti propositivi. E questo sta alla Presidenza constatarlo e darne atto. È stato e continuerà ad essere obiettivo principale di questa Presidenza... *(Brusìo in sto cercando di rispondere ad un garbato e importante intervento di un Capogruppo dell'opposizione e stiamo discutendo di un tema estremamente delicato. Presidente

non soltanto sulle affermazioni o sulle interviste, ma sui testi, dove si può realmente trovare un'intesa se vi è la possibilità di trovare punti di convergenza; e io sono fiducioso a questo riguardo. Sul calendario dei lavori lei

di non impegnare oggi l'Assemblea nell'esame di emendamenti, proprio perché occorreva dilatare correttamente il tempo per la presentazione di subemendamenti. Questo si è svolto nel solco del tentativo di conferire all'Aula sempre più dignità di spazio e sempre maggiore rispetto di quelle che sono le esigenze dei singoli parlamentari, sia di opposizione che di maggioranza, di poter esprimere le loro idee, perché la presentazione di un subemendamento - lei concorderà con me - è un diritto del singolo parlamentare al di là della sua appartenenza. E allora abbiamo deciso all'unanimità, con il solo voto contrario dell'Italia dei Valori (che non credo sia contrario su questa scelta, ma per le motivazioni da lei espresse),

l'impegno della Presidenza è stato, e sarà sempre, quello di fare in modo che la rappresentanza dei Gruppi sia garantita in tutti gli organismi interni al Parlamento. Questo è stato e continuerà ad essere l'auspicio di questa Presidenza, perché democrazia significa rappresentatività e rappresentatività significa avere la possibilità d'intervenire negli organismi che decidono le regole della vita interna del Senato.

postulerà forse una modifica del Regolamento ma, quando vi è la volontà, il Regolamento su queste tematiche credo si possa modificare in un batter d'occhio, in quanto la modifica è finalizzata a rendere rigorose le regole della corretta disciplina del voto.

di regole che migliorino la nostra qualità di vita parlamentare e la rendano più trasparente e più corretta. Noi siamo un Palazzo di vetro, siamo controllati e controllabili e rivendichiamo questa possibilità di controllo da parte dell'esterno. Sta a noi, con senso di responsabilità, trovare quei modi per lavorare meglio, per farci controllare meglio, per farci eventualmente criticare e recepire quelle critiche quando queste dovessero colpire anomalie di vita parlamentare che meritano di essere rivisitate e, eventualmente, anche corrette. Io non ho paura, come Presidente del Senato, di intervenire tutte le volte in cui dovessi riscontrare, così come ho fatto in passato, delle anomalie che vanno rimodulate, azzerate e cancellate. Dobbiamo guardare al domani, non al passato, non sarà il passato non sarà il passato il viatico del domani, almeno per quanto riguarda la gestione di questa Presidenza da parte del sottoscritto.

questo intervento sull'ordine dei lavori, anche se in effetti non è attinente all'ordine dei lavori, ma, poiché tocca un tema estremamente delicato, la Presidenza ha consentito al presidente D'Alia di svolgerlo. Attesa la delicatezza del tema, pregherei l'Assemblea

caso specifico perché possiamo renderci conto di che cosa stiamo parlando: «Auguri di buon anno, padrino Totò Riina, sei l'unico vero capo, il tuo carisma non ha ormai eguali»; «Bernardo Provenzano, forse a Natale si comincia subito con la beatificazione. Onore al re»;

composto da 422 iscritti, inneggia alla scarcerazione del noto mafioso. Qualche settimana prima, signor Presidente, lo stesso noto *social network* Facebook aveva ritenuto di non pubblicare non pubblicare foto di mamme che allattavano perché ritenute non consone allo spirito estetico e non solo estetico del sito stesso. Io non ho alcuna intenzione di discutere qui di questo *social network*, mi permetto solo di fare alcune brevissime riflessioni. Dopo che è scoppiata la polemica anche sugli organi d'informazione,

agli autori della strage di Erba, a Giovanni Brusca, a Pietro Maso, a Leoluca Bagarella. Ci troviamo dunque di fronte alla crescita esponenziale di un fenomeno

Inoltre, la Procura nazionale antimafia e la stessa Polizia postale in maniera assolutamente puntuale e precisa hanno dichiarato che il fenomeno non va sottovalutato, che è possibile che dietro questi *fan club* vi siano

di Facebook si sia limitato a dichiarare, in ordine a questa vicenda, che loro non hanno la possibilità per contratto di verificare l'ammissibilità dei profili. Cosa ci azzecca questo con la circostanza che siano state censurate le mamme? Che possano essere censurate le mamme e invece non vengano censurati le foto e chi inneggia a Toto Riina ci sembra quantomeno anomalo.

è anche quello di cancellarsi da Facebook qualora questi *fan club* non vengano cancellati. La ringrazio per la sua sensibilità.

la fine dei lavori, ma volevo solo augurarle buon anno anche da parte dei dipendenti dell'Alitalia che questo momento non lo hanno passato bene,

Auguriamo buon anno a tutti.

certamente da accogliere; anzi, vorrei aggiungere che domani, 14 gennaio, il gruppo «Fuori la mafia da Facebook» ha proclamato uno sciopero generale. Tutti coloro, parlamentari o meno, tutti i cittadini del mondo che vorranno protestare contro la mafia all'interno del *social network* Facebook, potranno farlo non accedendo alla propria pagina o al proprio *account*.

Su questo punto vorrei interrogare il Governo, così come ha fatto il senatore D'Alia, anche su altre questioni, certo meno gravi, come ad esempio la diffusione di siti *escort*, che sono abbastanza degradanti per i nostri giovani e per il genere umano. Pongo allora un quesito che credo sia alla base di tutto ciò: perché il fenomeno mafioso torna ad essere così penetrante nei giovani e viene inneggiato e addirittura individuato come soggetto referente e idolo della propria esistenza? Prima i giovani si incontravano in piazza o al muretto, mentre oggi si incontrano su Facebook: è una piazza. Allora la censura mi va bene,

la diffusione della cultura della legalità e uno stabile inserimento nel tessuto produttivo più virtuoso. Si tratta di un fenomeno complesso voglio apprezzare la proposta del senatore D'Alia di censura e di protesta, ma andrei ancora oltre, con degli interrogativi che forse ci dobbiamo porre.

Grazie, a conclusione di un dibattito che si è svolto alcune settimane fa e che ha riguardato un disegno di legge che lungo la strada

che riguardano la sicurezza ve ne sono alcuni sui quali si è lavorato con una buona intesa tra le forze politiche. Ad esempio, tutta la prima parte, che affronta il tema della sicurezza in senso lato, con aggravanti di pena per reati commessi in determinate circostanze

raggiunto un'intesa in materia di provvedimenti che renderanno sempre più intensa e forte la possibilità di combattere le mafie.

che ad avviso del tribunale di sorveglianza di Roma non è più un mafioso pericoloso e che ha potuto trascorrere tranquillamente il Capodanno a regime ordinario insieme a tutti gli altri carcerati per reati minori, probabilmente ricominciando da lì a intrattenere rapporti con il territorio per dimostrare che la mafia riesce a comandare anche quando è detenuta nelle patrie galere. Non è un caso che nel provvedimento al nostro esame vi sia un articolo che si occupa proprio del carcere duro, per inasprirne le condizioni, cercare di rendere molto più difficile la revoca, per creare un centro unico che prenda le decisioni, ma anche per regolamentare in modo diverso tutti i permessi carcerari, i comportamenti in carcere, le cose che i detenuti possono fare, assegnando pene molto più aspre di quelle attuali per i reati connessi alla comunicazione esterna. Vi è poi una parte che riguarda il codice della strada; anch'essa è stata oggetto di arricchimento nel dibattito in Commissione e negli emendamenti che sono presentati all'attenzione dell'Assemblea.

infingimenti. Ognuno di noi proviene da campagne elettorali nelle quali ha assunto impegni con gli elettori: quello che noi stiamo facendo è cercare di mantenere gli impegni assunti con gli elettori nel corso della campagna elettorale. Nessuno di noi si sogna un Paese chiuso ad esperienze che soggetti meno fortunati di altre Nazioni vogliono venire a fare in Italia, a patto che essi entrino avendo la possibilità di trovare un lavoro e non dovendosi procurare da vivere non lavorando e quindi

Chi deve lasciare l'Aula è pregato cortesemente di

cominciato ad uscire dall'Aula. Io stesso, come vede, sto replicando a braccio, dal momento che avevo lasciato l'intervento in ufficio pensando di doverlo fare domani mattina. Sono cose che capitano, ma l'importante è potervi fare fronte. Sulla parte che riguarda l'immigrazione ci sono certamente sono certamente contrasti ampi, ma dobbiamo venirne fuori in un dibattito sereno, con tesi diverse perché diversi sono gli impegni che abbiamo assunto con i nostri elettori, ma soprattutto - io credo - con la convinzione che nel nostro Paese si possa e si debba entrare,

lavorare. Chi vuole entrare nel nostro Paese deve sapere che dovrà rispettare le regole di convivenza civile, le leggi di questo Stato ed essere cittadino tra i cittadini, assoggettandosi a diritti e doveri e non pensando di poter reclamare soltanto diritti. Su questo il dibattito è aperto; ci sono visioni diverse ed emendamenti su cui

come il dibattito sia stato proficuo, come siano emerse una serie di indicazioni che possono essere sicuramente prese in considerazione e come anche il confronto tra maggioranza e Governo sia stato dialettico, consentendo anche a noi di apportare modifiche al provvedimento. Con queste considerazioni termino questa breve replica, avendo affidato la relazione ad un testo scritto che fa parte integrante del disegno di legge. Mi auguro che dall'esame dei molti emendamenti - circa circa 200 da esaminare - possa venire non un confronto su posizioni di maniera o solo per dimostrare che qualcuno ha presentato richieste di modifiche, ma un confronto di merito per cui se ci sono modifiche che possono essere accolte per migliorare il provvedimento, così come fatto in Commissione,

dal Parlamento; completiamo cioè un disegno più complessivo per fronteggiare i problemi dell'ordine e della sicurezza dei cittadini, impegno prioritario di questo Governo e della maggioranza: con questo passaggio stiamo onorando quest'impegno politico.

Signor Presidente, la discussione generale svoltasi nel mese di novembre ha sostanzialmente confermato la necessità avvertita dal Governo e dalla maggioranza di dare anche sul piano normativo una risposta efficace al problema della sicurezza pubblica e della criminalità, tanto di quella diffusa e apparentemente minore quanto di quella organizzata, che non può essere ridotto ad una mera questione di percezione da parte dell'opinione pubblica. Gran parte degli interventi, tanto di maggioranza quanto di opposizione, hanno infatti convenuto sulla necessità di un maggiore impegno dello Stato su questi fronti. Va osservato che anche nei diversi interventi dei colleghi dell'opposizione vi è stato un sostanziale riconoscimento della condivisibilità, almeno in linea generale, dell'approccio recato dal disegno di legge, legge, che da un lato ha tenuto conto anche di proposte prefigurate da un analogo intervento normativo a suo tempo predisposto dal Governo Prodi e, nel corso del dibattito in Commissione, di indicazioni e di suggerimenti provenienti dalla stessa opposizione. Ciò nondimeno, in alcuni interventi dei colleghi dell'opposizione sono state riproposte talune critiche su punti qualificanti del nuovo impianto normativo

dopo le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in particolare in materia di estensione del regime di reclusione previsto all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario a cui ha fatto prima riferimento il presidente Vizzini, secondo la quale il disegno di legge in titolo avrebbe espresso una filosofia della tutela della sicurezza pubblica eccessivamente sbilanciata nel senso della repressione della criminalità diffusa, definita come minore, rispetto all'impegno di un severo contrasto alla criminalità organizzata. Al contrario, occorre ribadire che il disegno di legge rappresenta senz'altro uno dei più significativi ed innovativi interventi degli ultimi anni in materia di elaborazione di strumenti giuridici utili a contrastare la criminalità organizzata e la sua infiltrazione nell'economia legale. Peraltro, anche gli interventi diretti a contrastare la criminalità cosiddetta minore vanno letti in un quadro organico, diretto a ripristinare l'autorità dello Stato e la sua capacità di presidiare tutti gli ambiti della vita associata. Ciò che non deve essere visto, come ha fatto ad esempio nel suo intervento il collega senatore Carofiglio, come l'espressione di una politica criminale cosiddetta di classe, diretta cioè a tutelare gli interessi dei gruppi sociali privilegiati nei confronti di quelli marginali, ma al contrario come il frutto della consapevolezza che sono i cittadini più poveri e deboli, (anziani, disabili, abitanti delle periferie) i più esposti alla criminalità diffusa, che proprio per la sua pervasività ed impunità finisce per contribuire in maniera significativa all'insicurezza e al degrado della vita di ampi strati della società italiana, così da non potere essere assolutamente qualificata come criminalità minore. Gli sforzi per ricondurre ad un organico e ordinato governo il fenomeno dell'immigrazione (contrastando la criminalità e quindi, per converso, anche la clandestinità), il tentativo di far emergere fenomeni per loro natura sfuggenti (quale quello del vagabondaggio) in maniera da metterli sotto il controllo dell'autorità pubblica, il contrasto a forme di sfruttamento odioso dei minori (come quelle legate al fenomeno dell'accattonaggio) e perfino la maggiore severità con cui si propone di affrontare l'imbrattamento ed il danneggiamento delle strade e dei palazzi delle nostre città non sono dunque fini a se stessi, ma sono diretti a restituire ai cittadini, in particolare proprio a quelli più deboli, il loro ambiente di vita e la possibilità quotidiana di poterlo vivere in serenità e sicurezza. In conclusione, pur nella consapevolezza che dal dibattito sugli emendamenti potranno venire ulteriori miglioramenti e perfezionamenti dell'articolato

pur non esaurendo la politica di contrasto alla criminalità e di sviluppo della sicurezza che il Governo sta perseguendo fin dall'inizio della legislatura, rappresenti certamente un momento importante per il ripristino nella società italiana di un clima di serenità e sicurezza, sempre auspicabile e che appare particolarmente necessario in un momento storico caratterizzato da una gravissima congiuntura economica mondiale, cui si potrà far fronte solo in un contesto di fiducia diffusa e di garanzia della sicurezza pubblica. Attendiamo su questi punti il contributo fattivo delle opposizioni.

hanno dato conto della completezza e dell'articolazione del dibattito, che interviene su uno degli aspetti fondamentali del complesso pacchetto sicurezza,

C'è, per esempio, la previsione del potere di accesso del prefetto in chiave di prevenzione antimafia nei cantieri; quindi, non soltanto quando già esistono rischi di infiltrazione mafiosa che si sono concretizzati, ma quando c'è il timore che si manifestino. Vi è poi una più incisiva possibilità di intervento sulle misure di prevenzione, soprattutto quelle patrimoniali, sancendo definitivamente la scissione tra la pericolosità personale e la provenienza mafiosa del bene. una chiarezza ed una trasparenza della figura dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati e poi confiscati, con la previsione di un albo nazionale cui si accede con precisi requisiti di competenza e di affidabilità personale.

143 viene riscritto non soltanto prevedendo clausole più chiare e precise, con ciò limitando quindifortemente la possibilità dell'impugnativa in sede di giustizia amministrativa ma anche integrando l'intervento dello Stato su una fascia che finora era rimasta esente dalla prevenzione antimafia, vale a dire non quella degli amministratori eletti ma quella della burocrazia degli enti territoriali. finora si è colpito il sindaco, l'assessore e il consigliere comunale ma non il tecnico comunale o il segretario generale, che in certi casi, in certe aree e in certi municipi, rappresentano l'elemento di continuità non della buona amministrazione

un mutamento non soltanto sul piano giuridico e politico ma anche su quello culturale in senso lato, è quella che sanziona l'inottemperanza all'obbligo di denuncia, raccogliendo l'esortazione

che omette di denunciare la richiesta estorsiva alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria compie un'attività che si avvicina a quella di chi gli rivolge la richiesta estorsiva che non a quella di una persona che vuole contrastare la mafia. Si è circoscritto il campo per evitare velleitarismi, colpendo lì dove effettivamente necessario, rispetto agli imprenditori aggiudicatari di una gara per l'esecuzione di lavori pubblici. In questo caso il meccanismo previsto è che al termine delle indagini il pubblico ministero che riscontra che vi è stata una richiesta estorsiva e che quest'ultima non è stata denunciata, rivolge rivolge una segnalazione all'autorità garante che a sua volta pubblica la segnalazione stessa sul sito; da ciò deriva un'interdizione dal poter ottenere appalti in futuro, oltre che una decadenza nell'appalto in corso. Ricordo poi le disposizioni richiamate dal presidente

di elementi in più per ricostruire flussi finanziari che finora sono rimasti nelle nebbie e che si muovono nell'area dell'illecito. Anche il Governo auspica,

"il paranoico direttore" che presenta stati di infermità mentale, quadri di delirio sistematizzato,un'azione coartata all'idea delirante che prevale, incapacità di intendere e di volere,

questo solo perché «il Giornale» in questi giorni ha ritenuto, seguendo una sua linea politica ed editoriale, di porre alcune domande - non so se esatte o no, ne porterà la responsabilità «il Giornale» - al senatore Di Pietro sulla gestione del patrimonio e dei contributi elettorali di quel partito. Credo sia davvero intollerabile che un senatore, un partito politico, un ex Sottosegretario del Governo Prodi si siano permessi di dichiarare delirante e paranoico il direttore di un quotidiano solo perché ha portato avanti una linea editoriale ed ha posto delle domande. Mi piacerebbe dire al senatore Li Gotti, come si diceva in un famoso film in cui recitava un famoso attore, «è la stampa, bellezza»;

solo perché scrive alcune cose su un libero quotidiano. Mi domando cosa sarebbe successo se cose di questo genere le avesse dichiarate un senatore di centrodestra su un direttore di un quotidiano di sinistra. Mi domando in quanti si sarebbero stracciati le vesti.

una compagnia che ha regalato solo cassa integrazione, licenziamenti e disperazione. Oggi non è nata una compagnia, ma una minicompagnia voluta da 16 persone, amici del presidente del Consiglio Berlusconi...

segnalato che molte famiglie, un indotto di circa 300.000 famiglie, non hanno festeggiato il nuovo anno: un 2009 fatto fatto sicuramente di tragedie poiché le famiglie non vedono più un futuro. Durante questi mesi i dipendenti Alitalia sono stati illusi, mortificati ed uccisi nelle loro speranze. Durante questi mesi, i 16 soci si sono impadroniti di Alitalia senza versare un euro. Collega Gramazio,

Alcuni di questi cosiddetti patrioti sono stati insigniti dal Capo dello Stato (fortunatamente non quello attuale) del titolo di Cavaliere del lavoro, che si riconosce a chi ha portato lustro ad un'azienda

il modo in cui è vestito in questo momento il senatore Pedica (che indossa il giubbotto degli operai di terra di Alitalia)

domani in quest'Aula a sostenere battaglie giuste, per esempio per gli uomini delle forze dell'ordine, vestiti da uomini delle forze dell'ordine che difendono la nostra libertà. Lei non può permettere ad un parlamentare

perché si veste in questo modo e partecipa a tutti i teatrini della burla politica che viene perpetrata ai danni dei lavoratori dell'Alitalia, a partire dal suo "capo", che è andato ad arringare, quando non ce n'era bisogno, i lavoratori di Alitalia. Quei lavoratori che sono stati salvati, perché se avessimo fatto quanto diceva o pensava

un uomo e un parlamentare che è travestito e non ha alcun rapporto con il mondo del lavoro dell'Alitalia.

Grazie, Presidente.

e a noi che rappresentiamo tanti di quei cittadini che in questo momento stanno iniziando a vivere gli effetti della pesante crisi economica

essa risultava scoperta (insomma, non coperta economicamente). So che lei si è attivato e che il Governo era anche disponibile a venire in Aula prima delle vacanze, ma poi la seduta

nei confronti di questo strumento, riguardo la verifica del suo funzionamento e del numero delle persone che effettivamente riescono a utilizzarlo.

elargire questi soldi direttamente su stipendi e pensioni, evitando questo inutile strumento propagandistico, che poi si sta prestando ai suddetti episodi. Quindi, al di là del fatto che - come dicevo - mi trovi nelle condizioni di doverle riproporre la questione,

Raccontava storie di emarginati, prostitute, drogati, criminali, soldati e suicidi, con grazia più che con sentimentalità. De André viene descritto come un uomo per molti versi contradditorio: *bohémien*, timido e sensibile, intellettuale e populista. Di ricca famiglia, era figlio del vicesindaco di Genova e per tutta per tutta la vita è stato anarchico. Lui e la moglie furono rapiti in Sardegna e tenuti prigionieri per quattro mesi. Dopo il rilascio mostrò scarso rancore verso i suoi rapitori, dicendo che erano prigionieri come lo era lui. aveva una conoscenza molto ampia; tradusse le canzoni di Bob Dylan e Leonard Cohen, scrisse canzoni insieme a grandi musicisti. Tuttavia, forse la ragione per cui De André rimane così celebrato è la sua spiritualità: cantava la condizione umana, parlava di amore e morte senza mai ricorrere a stereotipi; anche se ha sempre detto che trovava difficile credere in Dio, era pieno di ammirazione per Gesù e il suo album «La buona novella» si rifaceva ai Vangeli apocrifi; nonostante fosse al massimo un agnostico, De André scrisse canzoni che sembravano parabole ed oggi molte sono suonate perfino nelle chiese. Onorevoli colleghi, ringrazio la Presidenza per aver consentito

di ricordare in quest'Aula uno dei più grandi poeti del Novecento, un uomo libero e perciò osteggiato dal potere costituito che lo aveva persino schedato come sovversivo. *(Applausi Colleghi, riguardo all'intervento del senatore Bornacin, desidero dire che naturalmente la Presidenza non può e non vuole intervenire nella polemica politica, cioè non entra nella valutazione di un articolo, di un intervento

anche perché la Presidenza deve garantire il diritto di parlare in quest'Aula a chi è stato eletto. Per quanto riguarda l'intervento della senatrice Adamo, era stata già prevista un'informativa

il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha detto che se ne farà carico e comunicherà alla Presidenza del Senato quando si potrà svolgere

è al centro dell'attenzione, delle preoccupazioni, dei dubbi, delle domande di molti cittadini italiani. Infine, ringrazio il senatore